il Senato non è in numero legale

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 14 giugno. Come già previsto, oggi pomeriggio sarà anzitutto discussa la questione di urgenza relativa all'affare inerente la revisione delle leggi elettorali. Si passerà poi al seguito delle votazioni sul disegno di legge recante norme contro lo sfruttamento di lavoratori stranieri clandestini. Per consentire la partecipazione dei senatori alla Festa dell'Arma dei carabinieri, prevista questa sera, la seduta si concluderà entro le ore 18,30, auspicabilmente dopo l'approvazione del disegno di legge predetto. L'intera giornata di domani sarà dedicata alla discussione delle mozioni e degli altri documenti concernenti la vicenda vice ministro Visco-Guardia di finanza. Per le illustrazioni e la discussione generale - che avranno luogo dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,40 - sono state ripartite ripartite proporzionalmente tra i Gruppi sette ore. Alle ore 19,40 inizierà la trasmissione diretta televisiva della replica del Governo (venti minuti) e, a partire dalle ore 20, delle dichiarazioni dì voto dei Gruppi (dieci minuti ciascuno; quindici minuti al Gruppo Misto). Conclusa la diretta televisiva, sarà poi concesso un minuto a ciascun Gruppo per annunci di voto sui singoli strumenti da porre in votazione, come per prassi, secondo l'ordine di presentazione. Le votazioni avranno luogo indicativamente tra le ore 22 e le ore 22,30 di domani. Il disegno di legge recante delega sulla sicurezza sul lavoro è stato anticipato rispetto agli altri argomenti previsti dal calendario, e quindi anche rispetto al disegno di legge sulla liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, già all'ordine del giorno di oggi. Oltre alla delega sulla sicurezza sul lavoro, il calendario della prossima settimana prevede il decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania (a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 13 giugno), i disegni di legge relativi alla liberalizzazione dell'energia elettrica e del gas, al riordino dei servizi pubblici locali, nonché il disegno di legge comunitaria 2007.

sua decisione. La Commissione nazionale di garanzia ha censurato lo sciopero nazionale, indetto per il 16 e il 17 giugno prossimi,

Si tratta di uno sciopero indetto dall'Assemblea nazionale dei ferrovieri, organo di sindacato nato dopo il gravissimo incidente di Crevalcore, che attraversa tutte le sigle sindacali (dal sindacato extraconfederale a quello confederale) e che in questi anni ha proclamato diverse iniziative di mobilitazione e di lotta,

Il fatto che la Commissione di garanzia sostenga che i proponenti lo sciopero non siano

il ragionamento testé svolto dal collega, difendendo invece il ruolo della Commissione di garanzia per il diritto di sciopero, che ha sempre operato con estrema cautela e lo ha fatto anche in questo caso, nel momento in cui ha doverosamente constatato la mancanza di legittimazione nei soggetti che hanno promosso l'azione di sciopero.

il diritto di sciopero, da un lato, e il diritto degli utenti ad avere garantiti i servizi essenziali ed una minima continuità dei servizi stessi, dall'altro, si può ritenere essere si può ritenere essere stato nel nostro Paese regolarmente viziato con una maggiore tutela del diritto di sciopero e una minore tutela dei legittimi interessi degli utenti alla continuità del servizio. quindi che non sia giusto lasciare che una sola voce si rivolga alla Commissione di garanzia influenzandone impropriamente l'attività. Io aggiungo la mia voce di segno opposto affinché la Commissione, con ancora maggiore coraggio, raggiunga il punto di equilibrio fra gli interessi degli utenti e quelli dei lavoratori ad una legittima azione di sciopero. c'è da constatare come tutte le sanzioni promosse dalla Commissione di garanzia si siano sempre rivelate ineffettive. Tale ineffettività ha determinato sempre il conculcamento dei diritti dell'utenza,

dovremmo sempre rivolgerci, anche quando consideriamo il doveroso punto di equilibrio con l'altro interesse costituzionalmente tutelato, quello relativo al diritto di sciopero, che non viene in alcun modo leso, anzi. Mi sembra infatti che non si possa certo dire che in questo Paese vi sia, in alcuna misura, una limitazione del diritto di sciopero, che si esercita, come ho detto, anche in forme talora discutibili, prendendo in ostaggio gli utenti, nonostante la regolazione preveda

alla Guardia di finanza e al vice ministro Visco. Ci troveremo a discutere su alcune mozioni; nella nostra, che abbiamo integrato presentandola in una nuova versione, abbiamo sollevato il problema relativo alla mancata conoscenza degli atti di presunta revoca nei confronti del generale Speciale. Abbiamo lamentato il pericolo che ci si possa trovare, in questo momento e domani, dinanzi ad una situazione paradossale, cioè in presenza di un nuovo Comandante generale della Guardia di finanza, nominato con decreto del Consiglio dei ministri, sottoscritto dal Capo del Stato, che si andrebbe a sovrapporre ad altro Comandante generale della Guardia di finanza mai revocato. Ora, siccome non possiamo certo parlare di avvicendamento, tenuto conto che il generale Speciale non aveva raggiunto i limiti di età per poter essere dimissionato, trattandosi quindi di un atto sostanzialmente ablativo del suo *status*, occorreva un provvedimento esplicito attraverso il quale si significhino le motivazioni ed espressamente si affermi un principio inibitorio nei suoi confronti per la sua carica. Allora, prima ancora che domani si discuta di questo tema, noi, signor Presidente, vogliamo segnalare al Governo di fare preventivamente chiarezza sulla correttezza e sulla dinamica degli atti amministrativi che hanno portato allo sviluppo di questa vicenda. Si tratta - ripeto - di una situazione estremamente delicata; tra l'altro, nella storia della nostra Repubblica sono pochissimi i precedenti simili ed analoghi a quelli che si sono consumati nella giornata di venerdì. venerdì. Non vi è stato da parte del generale Speciale un consenso al suo dimissionamento; ha rinunziato ad accettare la sua collocazione presso la Corte dei conti. In conti. In passato, le sostituzioni potevano avvenire per via implicita perché poi si accompagnava il generale dimissionario ad altre cariche ovverosia non ve ne era bisogno in quanto, raggiungendo i limiti di età, non poteva proseguire nel suo incarico; ma tutte queste fattispecie sono diverse da quella che si è consumata venerdì. Credo allora che il Governo, essendosi assunta la responsabilità di compiere un atto di alta amministrazione (riteniamo che il provvedimento di venerdì rientri negli atti di alta amministrazione e non soltanto di scelta politica), sia tenuto a dare contezza al Parlamento della discrimina degli atti giuridici posti in essere. Chiediamo, quindi, al Governo di fare chiarezza, ancor prima del dibattito, perché non vorremmo che il Paese si trovasse in presenza

la richiesta che le faccio è determinata da un fatto accaduto in questi giorni: una multinazionale americana, che ha stabilimenti anche in Italia, oltre oltre che in America e in Cina, ha richiamato tutto il *management* italiano dagli stabilimenti cinesi in quanto, a detta loro, nel distretto di Shanghai è in corso un'epidemia di tifo.

chiede di conoscere l'entità del fenomeno e di avere quanto prima il nostro Ministro della salute al Senato per illustrare cosa sta accadendo, dal momento che i traffici tra Italia e Cina,

sollecitare, sottoponendola alla sua attenzione, un'interrogazione che ho presentato oggi riguardante i fatti accaduti a L'Aquila i fatti accaduti a L'Aquila domenica scorsa, dove vi è stato un corteo di manifestanti sotto il carcere di massima sicurezza, nel quale è ristretta

che si verifica in questi ultimi tempi. Si tratta di un fenomeno inquietante: la diffusione del messaggio brigatista è arrivata ad una forma tale di spavalderia da manifestarsi anche nei cortei in maniera così evidente, senza alcuna forma di segretezza, tipica

per lo Stato. Chiedo che su questi temi il Ministro dell'interno intervenga al più presto, anche perché in settimana vi sarà la visita del presidente Bush e non vorrei che queste manifestazioni fossero preparatorie di manifestazioni ben più gravi di «accoglienza» al Presidente di un grande alleato dell'Italia, gli Stati Uniti d'America. Presidente, un'ultima battuta sul tema sollevato dal Presidente del mio Gruppo. La questione posta dal presidente Schifani non si può discutere domani: dev'essere risolta entro domani, perché ci troveremmo di fronte a una vicenda paradossale, dove non vi è un provvedimento di alta amministrazione, espresso nelle forme di rito, regolato dalla legge, sottoscritto dal Presidente del Consiglio, deliberato dal Consiglio dei ministri e controfirmato dal Presidente della Repubblica,

in secondo luogo, perché essa non può intervenire per annullare una dichiarazione di sciopero del tutto conforme alle norme di autoregolamentazione e alla normativa di legge. Esprimo ulteriore preoccupazione perché avevo avuto modo di segnalare ai Presidenti di Camera e Senato come la composizione

preoccupante che il pronunciamento della Commissione di garanzia si collochi a valle di una decisione già discutibile del Ministro, che ha ritenuto di dover ridurre a otto ore lo sciopero proclamato dai sindacati confederali, e di una dichiarazione, francamente inaccettabile, dell'amministratore delegato delle Ferrovie

di rilievo e tempi fissati da una scadenza, quella della festa dell'Arma dei carabinieri, a cui tradizionalmente deputati e senatori sono interessati.

sollecitare a lei la discussione del primo punto all'ordine del giorno: trattandosi di un'urgenza, non vorremmo che oltre la melina ci fosse anche un ostruzionismo rispetto all'urgenza. PRESIDENTE. Ma la melina diventa generale, poi, è un esempio contagioso, senatore Calderoli. Negli alberi di mele dopo una mela ne viene sempre un'altra, signor Presidente. In secondo luogo, visto che l'argomento sollecitato dal senatore Schifani è oggetto di strumenti di sindacato ispettivo e di ordini del giorno da parte del nostro Gruppo, francamente, Presidente, le chiedo, nel caso in cui non dovesse venire pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto di nomina (e credo che i passaggi che hanno preceduto tutto questo abbiano da una parte una celerità sospetta, dall'altra un mancato riscontro cartaceo), che la

convenga con la Costituzione.

lo abbia ripreso. Lei, signor Presidente, molto correttamente, ha detto: la questione domani è all'ordine del giorno, ne discuteremo domani. Ma noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di presentare documenti: e come facciamo, allo stato, a presentarli? In questo modo la mozione che è stata sottoscritta da tutti

si è preso atto della dichiarazione di Visco che rinunciava alla delega sulla Guardia di finanza e si è provveduto a deliberare l'avvicendamento. prima considerazione da fare: questo avvicendamento, sotto il profilo istituzionale, è corretto? E, soprattutto, ci sono state le motivazioni così come prevede la legge? Infatti, se non ci sono state le motivazioni,

e di nominare al suo posto altro generale, ma non si è provveduto a questo perché il generale alla Corte dei conti non è andato, allo stato, come rimarcava il collega Calderoli, ci sono due

Bisogna che il Governo questa sera, e non domattina, chiarisca questo aspetto, in modo da mettere in condizione non soltanto i Gruppi dell'opposizione, ma anche quelli della maggioranza, di scrivere documenti secondo quello che è accaduto. La confusione che si è determinata in queste ore dal punto di vista giornalistico ci interessa relativamente, ovvero ci può interessare come interessa ad ognuno di noi che ha deciso di fare questo mestiere, nell'Aula parlamentare abbiamo bisogno di sapere di cosa discuteremo domani per presentare un documento (una mozione, un ordine del giorno, un documento di sindacato ispettivo) che tenga conto di quella che è la situazione reale, perché allo stato si è determinata una confusione tale per cui non riusciamo a capire.

è stato vivacemente, ma civilmente, contestato da una rappresentanza dei movimenti di Vicenza per la vicenda dell'allargamento della base USA. la protesta della cittadina di Vicenza, rappresentata appunto in quei movimenti, non è stata trasmessa dal TG1 in *real* *audio*, come avrebbe dovuto essere, ma attraverso un'informazione manipolata

Io ritengo che il ruolo del servizio pubblico sia quello di assicurare un'informazione corretta e trasparente e non un'informazione manipolata. Tutto ciò è molto grave. Signor Presidente, noi chiediamo un suo intervento affinché il direttore del TG1 sia più rispettoso della verità

quell'occasione abbia assunto un solenne impegno, quello di ricordare gli agenti di polizia e gli uomini di legge che cadono per mano dell'eversione e del terrorismo. Domenica a L'Aquila uno degli *slogan* principali di duecento terroristi organizzati che hanno manifestato per le vie della città era:

sollecitato il prefetto e il questore di L'Aquila a vietare quella manifestazione in cui si gridava anche: «Biagi ora non pedala più».

dove sono stati sparati razzi e lanciati oggetti contundenti nei riguardi delle forze dell'ordine. E mentre si svolgeva questa manifestazione all'esterno, coloro i quali erano in carcere hanno sventolato dalle finestre dell'edificio bandiere rosse e gridato *slogan*.

Ci stiamo poi apprestando a ricevere il presidente Bush, ma non è questo il problema. Il problema è che i siti *web* e tutti quelli dell'ultrasinistra avevano annunciato

nel più breve tempo possibile, il vice ministro Minniti o il Ministro dell'interno per rispondere ad una serie di interrogazioni che riguardano gli atti di terrorismo concreto che si sono verificati domenica nella città di L'Aquila.

della discussione per evitare di trascorrere il tempo delle nostre sedute discutendo di argomenti che non sono all'ordine del giorno. Presidente, vorrei sottolineare che i diritti dei colleghi a chiedere la parola e ad ottenerla, in questa fase dei nostri lavori, sono disciplinati dall'articolo 84 del Regolamento, al comma Questo comma recita testualmente: «Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti». Questo è un diritto che viene esaminato dalla Presidenza nei modi in cui stabilisce il Regolamento. In questo caso, Presidente, io ho chiesto la parola ai sensi dell'articolo 92, che è un altro articolo articolo che disciplina i nostri lavori e che dice che i richiami al Regolamento - cosa che sto facendo o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza su tutto. Quindi, mentre gli interventi di questo tenore e di questo contenuto hanno la precedenza, quelli per i quali si intende discutere di un argomento non previsto all'ordine del giorno sono rimessi alla discrezionalità della Presidenza. la Presidenza del Senato, sia quando presiede lei, ma anche quando presiedono i Vice presidenti, è molto larga e comprensiva e consente a tutti di parlare, e francamente io sono anche favorevole;

non si farebbe più niente. Alla luce di ciò, vorrei soltanto chiederle di usare *cum grano salis* questo potere discrezionale della Presidenza,

cercare di contemperare tutte le esigenze, in maniera che si possa anche ogni tanto votare sulle questioni all'ordine del giorno.

tra le tante questioni che il Paese legittimamente discute c'è anche la questione della funzionalità e della capacità delle Aule parlamentari ad affrontare i problemi di merito. Poiché questo è un punto che aleggia nella vita e nel dibattito del nostro Paese, mi rivolgo a tutti i parlamentari, di una parte e dall'altra, perché accanto all'esercizio di diritti sanciti dal Regolamento ci sia anche la possibilità di rendere produttive le sedute della nostra Camera.

si sia rifiutato di accettare la rimozione e purtroppo in quel Paese allora la cosa è finita nel sangue. Il problema non può esistere in Italia perché la serietà, l'impegno e la dedizione della Guardia di finanza fanno sì che quei finanziari obbediranno al generale che è stato legalmente nominato. Dunque, esiste un solo comandante, l'altro è illegale e va bene per le

intervengo per un richiamo al Regolamento sulla questione posta dal collega Boccia e le assicuro che non replicherò alle sciocchezze dette dal senatore Colombo: la diretta televisiva ci sarebbe voluta adesso per far capire all'Italia che gente abbiamo di fronte!

Allora, vorrei poter parlare come si conviene in un'Aula del Parlamento. Signor Presidente, vorrei che fosse fissato un punto di chiarezza da parte sua e condivido appieno la sua osservazione rispetto all'intervento del senatore Boccia

84; però, non prenderei per oro colato la tesi che qui si è sforzato di sostenere, soprattutto perché ci sono precedenti numerosi di ostruzionismo che non mi sono dimenticato:

Il Presidente del mio Gruppo ha detto una cosa molta semplice: qui c'è il Ministro per i rapporti con il Parlamento, vogliamo sapere se quello che è stato denunciato prima dal presidente Schifani e poi dal presidente Matteoli è vero o non è vero, se c'è stata una deliberazione per scrivere una mozione secondo i nostri intendimenti,

sull'attuazione dell'articolo 92 del Regolamento. Resta inteso che, di fronte alla richiesta avanzata dal Gruppo parlamentare cui mi onoro di appartenere, mi aspetterei da parte del Governo un chiarimento, in modo che il dibattito di domani possa svolgersi secondo i crismi della correttezza parlamentare.

di cui mi compiaccio), significa che in questo momento la Guardia di finanza non ha alcun Comandante generale. Ma credo che questa situazione non sposti

il collega Colombo ha espresso delle parole di offesa nei confronti di un galantuomo, credo che l'Assemblea debba delle scuse ad una persona persona dichiarata illegittima nella sua carica. Il generale Speciale è un galantuomo, è ancora generale della Guardia di finanza e credo che il Senato, nella sua unanimità, debba delle scuse alle offese che se gli sono state profferite. *(Applausi dai

trovare, anche da parte del Presidente del Senato, una sollecitazione in queste ore, perché anche il sottoscritto, per la buona conduzione di un dibattito che domani

una dichiarazione, riportata tra virgolette, del generale Speciale che vorrei rendere nota all'Aula, perché mi sembra importante in questo momento. Il generale Speciale afferma: «Il Governo legittimo della mia amata Repubblica ha adottato nei miei confronti un provvedimento che io accetto, rettificando la posizione, mettendomi sull'attenti e dicendo semplicemente: "Obbedisco"». Credo sia una dichiarazione importante per l'Assemblea e per i nostri lavori. STORACE

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti. non più di dieci minuti. Seguirà poi la votazione per alzata di mano. Ha chiesto di parlare il senatore Calderoli per illustrare la sua richiesta di dichiarazione d'urgenza.

Riconosco la paternità della definizione e non di una legge che voleva essere una legge proporzionale con premio di maggioranza e che, nel corso dell'esame in Parlamento, ha subito modifiche che hanno portato ad evidenziare alcuni limiti oggettivi, in ragione soprattutto della possibilità di una governabilità del Paese, con un premio di maggioranza, attribuito a livello regionale al Senato, che fa emergere maggioranze casuali non certo idonee per la governabilità del Paese (i famosi «listoni bloccati», i famosi «sbarramenti» che tali non sono) e la possibilità di ogni partito, anche nell'ordine dei 10.000 voti, di poter concorrere per la definizione di una maggioranza. Oggi è in corso - anche qui, fuori di Palazzo Madama - una raccolta firme per un *referendum* che, a parole, vorrebbe andare verso il bipolarismo e una maggiore governabilità. Purtroppo - forse non sarà nelle intenzioni dei referendari - ma, di fatto, si realizzerebbe un qualcosa che è addirittura peggio del «*Porcellum*», perché non solo la governabilità non verrebbe garantita, visto che il premio

quel premio di maggioranza, paradossalmente potrebbe ottenerlo con un voto in più, raggiungendo il 55 per cento della maggioranza in seno al Parlamento. Credo che si debba ritornare alla legge Acerbo per trovare qualcosa di così antidemocratico! Oltre a non garantire la governabilità, si elimina il distacco tra l'elettore e l'eletto perché non ci saranno tante liste di partito, bensì un'unica lista, dove un'unica persona deciderà chi saranno gli eletti del centro-destra e chi del centro-sinistra. Probabilmente, al Senato non ci sarà un'unica lista ma, visti gli sbarramenti regionali, avremo cinque coalizioni che si presenteranno e pertanto la maggioranza la si costituirà dopo il voto, come ai bei tempi della Prima Repubblica. non è in grado di garantire la governabilità e la stabilità di Governo, mette a rischio la rappresentatività democratica di forze politiche fortemente radicate sul territorio o di forze politiche che qualcuno chiama «i partiti minori». Ma non è colpa dei partiti minori se 12 milioni di italiani votano quelle forze politiche: questa è la democrazia. E se qualcuno pensa, attraverso un *referendum* o per legge, di fare quello che non si è realizzato nella testa del Paese e neanche nella classe politica, ovvero di realizzare un partito unico del centro-destra e del centro-sinistra, mi spiace, ma si fa una «porcata» all'ennesima potenza. oggi, visto che abbiamo ancora lo spazio per poter far legiferare il Parlamento rispetto a questa materia, credo che debba esservi un'assunzione di responsabilità. Giacciono in Commissione, credo ormai più di dieci progetti di legge in materia elettorale e personalmente ne ho presentato uno per l'abrogazione della legge attuale e la rientrata in vigore del cosiddetto Mattarellum ed uno che si richiama al cosiddetto *Tatarellum* delle elezioni regionali con alcune integrazioni anche per poter riavvicinare il popolo alla politica. Personalmente, son convinto che non siano le leggi elettorali a risolvere la crisi della politica e i costi della politica e che tanto possa essere realizzato anche a livello di Regolamenti parlamentari. Io avrei presentato un ordine del giorno; l'articolo 77 non me lo consente, credo che da quest'Aula debba venire un forte impegno rispetto alla Giunta per il Regolamento per rivedere tutti quegli articoli che fino ad oggi non hanno consentito di contrastare la frammentazione politica, la proliferazione e la nascita di partiti fasulli, fasulli, perché non è possibile pensare che chi viene eletto in una lista, il giorno dopo costituisca una lista da un'altra parte! Questa è la libertà del mandato, ma non è lecito pensare che trasferimenti economici di beni e servizi vengano garantiti dal Senato anche a chi ha tradito il proprio elettorato. Ne vediamo un esempio tutti i giorni. Ci sono riforme costituzionali da completare: ben vengano, sono le stesse che abbiamo approvato nella passata legislatura. La nostra legge, proprio perché i tempi delle riforme sono diversi, prevede l'applicabilità del provvedimento sia a Costituzione vigente, sia a Costituzione variata, cioè nel caso fosse ridotto - come tutti auspicano - il numero dei parlamentari e fossero modificate le funzioni di Camera e Senato. Oggi non è

momento che chiaramente il Presidente della Repubblica ha indicato che non si può andare al voto con l'attuale legge elettorale, o si abroga la legge attuale oppure se ne scrive una nuova, assumendoci le nostre responsabilità. Se non lo si vuole fare e si vuole dar corso al *referendum*, significa che il Parlamento vuole abdicare alla propria funzione legislativa. Ma quando la ragion d'essere di una Camera viene meno, allora è meglio che venga meno la ragione d'essere della Camera. *(Applausi

colleghi senatori, la votazione odierna risponde ad una precisa responsabilità, ovvero dar vita ad una legge elettorale che consenta ai cittadini di sentirsi nuovamente rappresentati dalla classe politica. Opportuna è quindi la scelta di accelerare la discussione della riforma, dimezzandone - come previsto dall'articolo 77 del Regolamento - i tempi procedurali. La materia non è di quelle su cui il Parlamento ed il Governo possono permettersi d'indugiare oltre, persistendo in un limbo decisionale letale per la democrazia: letale poiché incombe come la spada di Damocle sul Parlamento il *referendum* Segni-Guzzetta. Tutti noi, infatti, sentiamo forte la necessità di archiviare l'*empasse* istituzionale di questi mesi per superare, con condiviso sforzo, la normativa vigente. In breve, occorre puntare ad un faccia ad un faccia a faccia tra i partiti, guidati dal dovere di costruire una legge elettorale che non pregiudichi politica e democrazia e, sopra ogni altra valutazione, i cittadini che rappresentiamo. Nel cammino di riforma, comunque, sarà puntuale il monito dell'Udeur (e non solo) a mantenere sempre fermo il duplice obiettivo di preservare la rappresentatività e la governabilità delle istituzioni in un sistema bipolare che garantisca stabilità e coesione delle coalizioni. Il *referendum* elettorale Guzzetta-Segni mina proprio il criterio della coalizione e riduce l'ipotesi bipolare ad un'ipotesi bipartitica secondo un criterio di convenienza che tocca a destra e a sinistra alcuni partiti a scapito di altri. Unico effetto del *referendum*, infatti, sarebbe la spaccatura in due del sistema politico italiano con la conseguente messa al bando dei partiti minori. È infatti in corso una campagna tendente a convincere i cittadini che il problema della governabilità si risolverebbe con l'annientamento dei piccoli partiti. Non si considera invece che sarebbe ben possibile confrontarsi su ipotesi di riforma della legge elettorale tali da conciliare governabilità e rappresentatività, considerando in modo differenziato le formazioni politiche minori, dando cioè spazio a quei partiti che hanno un forte e consistente radicamento in alcuni territori del Paese, che danno voce effettivamente alle realtà di riferimento. Siamo tutti concordi sull'opportunità di cambiare l'attuale sistema elettorale, che ingabbia la politica nella logica dei potentati forti ed annulla l'interclassismo, ma intendo in questa sede ribadire il fermo no del Campanile al *referendum* liberticida Guzzetta-Segni ed ai tentativi più o meno celati degli squali di mangiare i pesci piccoli: inconcepibile sarebbe una fauna marina fatta solo di squali! La reale alternativa al *referendum* ed ai summenzionati tentativi di cancellazione dei piccoli partiti a forte vocazione territoriale è quella di arrivare, con serena discussione aprendo il dialogo ed il confronto tra tutte le forze politiche, ad una legge elettorale che sia definitiva, idonea a ripristinare il contatto tra gli elettori e gli eletti, nonché a garantire la maggioranza alla coalizione vincente. Concludendo, devo ribadire la forte e tempestiva necessità che investe il sistema politico a rinnovare se stesso e nel contempo devo esortare ad avere il coraggio di cambiare. Occorre, cioè, dare il via alle riforme istituzionali ed *in primis* a quella elettorale, fissando le regole insieme, senza ricatti e senza imporre una volontà prevaricatrice e sorda alla voce dei partiti minori. Questi, dunque, sono i motivi del mio voto sull'urgenza della riforma elettorale. *(Applausi del

vi è l'esigenza che sulla legge elettorale sia il Parlamento, con un ampio schieramento, a dotarsi di una nuova legge. una nuova legge. È opinione comune ed unanime di tutti i partiti che l'attuale legge elettorale

In primo luogo, un partito, nel caso si presentassero almeno quattro liste elettorali e quattro partiti,

a collocarsi all'interno di un'unica lista, rispetto alla quale decide il capo - alla faccia della democrazia e della verifica elettorale, poi, dei parlamentari!

anche la cosiddetta bozza Chiti, che non è un disegno di legge, ma l'illustrazione di alcuni princìpi che sono il comune il comune denominatore delle consultazioni che il Ministro ha condotto a nome della Presidenza del Consiglio e che quindi raccolgono

che assuma il criterio fondamentale della larga rappresentatività del Parlamento, quindi delle idee e delle opinioni che ci sono all'interno della nostra collettività nazionale, e che si ispiri

ad adeguarsi, ad una legge elettorale che, per soddisfare le esigenze della semplificazione politica e della governabilità, si proponesse l'obiettivo della cancellazione di tutte le forze minori.

sia parlamentare in termini di voti, all'interno di questo ramo del Parlamento come nell'altro. *(Applausi

al di là dello scetticismo che su questa materia ho avuto modo di manifestare nel corso dell'intero anno che ci separa dalle ultime elezioni. Faccio, infatti, parte di quelli che non credono si procederà presto ad alcuna legge elettorale. Mi auguro che i colleghi che voteranno a favore della procedura d'urgenza, giustamente chiesta dal collega Calderoli, si impegnino seriamente a cercare di predisporre presto elettorale. Il mio scetticismo si basa su due questioni di fondo: non ho mai creduto alla possibilità di distinguere e di separare il dibattito e la deliberazione su una legge elettorale da quelli sulla riforma costituzionale: il Presidente della Camera e il Presidente del Senato hanno ripartito i compiti tra le due Assemblee in un modo apparentemente corretto, ma che, dal punto di vista sostanziale, rende di fatto impossibile qualunque riforma costituzionale, senza pensare anche ad una parallela legge elettorale o ad una riforma elettorale, senza sapere a quale sistema costituzionale si dà vita.

anche esaminando la storia della nostra Repubblica, non aver presente il fatto che il Parlamento non ha mai approvato una legge elettorale, se non a maggioranza politica: quando è stata elaborata una legge elettorale dopo il *referendum,* si è trattato di una legge elettorale di fatto imposta dal voto popolare a maggioranza popolare.

Come si può non aver presente che quella legge elettorale è tale proprio perché è prevista l'elezione diretta del Presidente della Regione e che non avrebbe senso una legge elettorale nazionale per eleggere

Dopo otto mesi di dibattito su questa vicenda, non è pensabile che si possa continuare a ritenere di adottare il sistema elettorale regionale, facendo finta di non sapere che esso è figlio di una legge elettorale che prevede un sistema costituzionale diverso da quello nazionale, a meno che non si dica

Avrei pertanto avuto piacere se in questo dibattito sulla procedura d'urgenza si fosse almeno sgomberato il campo da considerazioni che rendono impensabile la produzione legislativa di una qualunque legge elettorale.

eravamo giunti alla soppressione del cosiddetto bicameralismo perfetto e siamo stati sommersi da ogni tipo di critiche. Vorrei capire se stiamo parlando della stessa cosa. Se

Se vogliamo seriamente parlarne, ritengo che l'opinione originariamente indicata dal Ministro vada ripresa. Occorre che le due Camere deliberino un atto di indirizzo politico-costituzionale che faccia capire se si intende mantenere l'assetto costituzionale esistente, se vogliamo modificare la legge costituzionale riguardo al Governo, e in che modo, e quindi se vogliamo una legge elettorale che preveda una o due Camere. Quando avremo approvato un atto di indirizzo politico di questo tipo, allora potremo seriamente dire in quanto tempo - probabilmente poco - potremo fare una legge elettorale, ma non vedo nessun orientamento in questo senso. La stessa procedura d'urgenza indicata dal collega Calderoli non è ancorata a tale premessa, che in questo momento faccio come offerta al dibattito. dire al Presidente del Senato e al ministro Chiti che avrei molto piacere, come Capogruppo dell'UDC, se in un tempo molto rapido, intendo dire poche settimane, pochi giorni da oggi, vi fosse un atto di indirizzo politico‑costituzionale di entrambe le Camere, non soltanto del Senato della Repubblica, che ci faccia capire su queste tre questioni preliminari dove andiamo a parare. Anche perché vorrei che si uscisse da un generico parlare di legge elettorale, soprattutto dai colleghi rappresentanti dei cosiddetti partiti minori. Vengo alla questione dello sbarramento. Qui occorre chiarire se condividiamo l'opinione, largamente diffusa nei mezzi di informazione, che la frantumazione politica in molti partiti, presenti in Parlamento con numeri esigui di rappresentanza popolare, è un problema della democrazia. Non Non è infatti possibile immaginare che lo sbarramento di per sé sia il bene e il mancato sbarramento di per sé sia il male. Occorre capire se i rappresentanti di partiti minori ritengono di voler procedere (per via politica, non per via legislativa) ad aggregazioni politiche, immagino omogenee dal punto di vista degli obiettivi, e in tal caso essere pronti anche ad una legge elettorale che dia per presupposto che i partiti presenti in Parlamento non siano più tanto numerosi. Ma se così non è, di quale sbarramento intendiamo parlare? Lo dico, perché anche il mio partito ha ripetutamente indicato la preferenza per un modello ispirato a quello tedesco,

era divisa in due Stati, in uno dei quali era presente il partito comunista tedesco. Era molto facile avere uno sbarramento avendo risolto per via istituzionale il problema del partito comunista in un altro Stato: quello sbarramento aveva un senso che finiva con l'essere quasi esclusivamente sul versante della destra. Occorre capire, in altri termini, se parliamo di uno sbarramento perché vogliamo per così dire impedire la presenza di una pluralità di forze politiche nella sinistra del nostro Paese, oppure lo vogliamo perché vogliamo impedire un numero elevato di partiti. Di tali questioni abbiamo mai seriamente parlato nel Parlamento della Repubblica? Ritengo di no. Ecco perché, signor Presidente, insisto nel dire che il Gruppo è favorevole all'accelerazione della procedura, ma poniamo due esigenze: la prima, che ci sia un voto politico impegnativo in entrambe le Camere (Camera e Senato) sulla questione dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, se cioè esso sia ancora basato su due Camere o no, e ove sia basato su una Camera indicando il tipo di Camera che vogliamo avere (delle autonomie, delle Regioni, del federalismo, del secondo grado, ancora non ho capito di cosa si deve parlare, non pretendo un disegno di legge concreto); la seconda, se vogliamo una forma di Governo ancora parlamentare, con un Governo che ha bisogno della fiducia o meno, e quindi di quale legge elettorale parliamo. Con una precisazione, e mi rivolgo ai colleghi di qualunque Gruppo: vi siete chiesti perché in nessuna parte d'Europa esiste il premio di maggioranza? Vi siete chiesti, sulla questione del premio di maggioranza che viene dato per acquisito, qualunque sia la maggioranza ottenuta

politica di fondo che impedisce ad una maggioranza popolare o, meglio, ad un voto popolare non di maggioranza di diventare maggioranza parlamentare? Vogliamo capire che sarebbe inimmaginabile avere una maggioranza parlamentare ampia a fronte di una minoranza popolare risicata o addirittura risicatissima?

e la subordino alla seguente condizione politica: che si proceda in tempi rapidi a capire se abbiamo seriamente intenzione di procedere a questa riforma o se continuiamo a fare finta di volerla. Temo che nel Parlamento i deputati e i senatori eletti con questa legge elettorale avranno una difficoltà drammatica a passare ad una legge elettorale nella quale non vi è più la garanzia della rielezione per nessuno. *(Applausi

che riguarda il licenziamento dell'ex direttore dell'ANSA Magnaschi. L'interpellanza è stata presentata oggi, ma lei si renderà senz'altro conto che in questo caso sarebbe

La seduta è tolta